L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

quindi, di fatto, è stata impedita l'illustrazione degli ordini del giorno. Questo provvedimento si sta trascinando a singhiozzo in Aula:

Anzitutto, credo sia utile la lettura di questo primo ordine del giorno, perché con un parere contrario del relatore e del Governo in realtà si fa un'altra operazione, che è quella di dire che al relatore

Il Senato, premesso che: la proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense (CNF), rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e seguenti e articolo 32 e seguenti del disegno di legge); considerato che: siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private, che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati, impegna il Governo: - a provvedere a modificare il testo eliminando la previsione di un'attribuzione di potestà regolatoria in

si affida al Consiglio nazionale forense un triplice ruolo: innanzitutto quello di legislatore, e non solo come artefice del codice deontologico, che per la Cassazione, lo ricordo, ha forza di legge, ma anche come integratore attraverso una marea di regolamenti regolamenti delle lacunose norme di legge; poi, gli si affida anche il compito di amministratore: i poteri del CNF nei confronti dell'Ordine degli avvocati, con conseguente mostruosa carenza di terzietà del Consiglio nazionale forense quando sia vestito da giudice negli atti posti in essere in tema di disciplina e tenuta degli albi, da quei medesimi ordini locali dei quali il CNF

3, dove si prevede, al comma 3, che le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono ancora tutte emanate dal Consiglio nazionale forense,

È ancora peggio quando agli articoli 32 e 33 si definisce il Consiglio nazionale forense.

le pagine dei giornali di stamani sono piene di quanto detto dal Presidente della Repubblica ieri nell'incontrare i nuovi magistrati: in sostanza, si chiede ai magistrati di fare autocritica. autocritica. Non è che da questi banchi si possa chiedere all'avvocatura di fare autocritica, però, in base a quanto ci è stato detto, questa proposta è stata ampiamente condivisa con l'avvocatura italiana nel merito e anche nel metodo, dando adito a critiche molto aspre che hanno occupato parte della nostra discussione generale relativamente al fatto che risulta poco liberale (non che all'interno della maggioranza vi siano, ahinoi, esempi fulgidi di questa ideologia politica) coinvolgere gli interessati ad autoriformarsi, perché in effetti il rischio che venga fuori tutto tranne che una riforma è altissimo. Questo secondo ordine del giorno, sottoscritto dalle senatrici Poretti, Bonino e dai senatori Ichino, Sangalli e da me, affronta la questione, anch'essa sollevata dall'*Antitrust,* relativa all'accesso alla professione. Noi riteniamo che questa proposta di governo della professione forense tutto sia tranne che qualcosa in linea con una società aperta alla concorrenza, all'accesso alle professioni ed alle critiche, visto e considerato che purtroppo, anche su questo ordine del giorno, che ancora una volta recepisce le critiche dell'*Antitrust*, tanto il relatore quanto il Governo hanno dato un parere negativo. dai rappresentanti della professione liberale - che non necessariamente, ripeto, devono essere liberali, ma che tuttavia hanno a che fare con il rispetto dei diritti - preoccupa. Leggo le parti che secondo noi sono salienti. Si ricorda cioè ancora una volta il parere dell'*Antitrust*, dove si rileva che le nuove misure relative all'accesso alla professione forense, previste nel disegno di legge in esame, esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio e limitando in tal modo la flessibilità dell'aspirante avvocato che, in una fase del tutto prodromica e densa di incertezze rispetto al momento dell'effettivo inizio dell'attività con il conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense (articoli 40 - 42 del disegno di legge); l'*Antitrust* aveva inoltre osservato «che l'iscrizione al registro dei praticanti, per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, secondo quanto previsto nel di legge in esame, viene subordinata al superamento di un *test* di ingresso». Questo tipo di tecniche ha dato ampia dimostrazione di essere inefficace in altri contesti. Numerose sono le nuove limitazioni relative all'attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, con l'esercizio dell'attività di impresa e con lo svolgimento anche di altri tirocini; viene inoltre limitato l'ambito di attività professionale proprio del tirocinante, prevedendo così che lo stesso, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale iscrivendosi all'Albo dei praticanti abilitati al patrocinio, ma soltanto in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità. Questa disciplina, dal punto di vista concorrenziale, secondo l'*Antitrust* ma anche secondo chi avrebbe incluso all'interno del proprio programma di Governo un punto fondamentale, la libertà di mercato mirando ad eliminare quanti più limiti possibili all'irrigidimento tipico e burocratico di un settore economico italiano, irrigidimenti ed impedimenti burocratici che per l'appunto, nella scorsa legislatura, il Governo Prodi, grazie all'allora ministro Bersani aveva iniziato ad allentare), appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche degli avvocati abilitati, che possono avvalersi dell'attività dei tirocinanti eventualmente a titolo gratuito, e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel codice deontologico degli avvocati, dove, all'articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo un periodo iniziale, l'avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Non contemplare nella proposta di riforma una disposizione di analoga portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della semplice possibilità di svolgere la pratica forense. In sede di replica il relatore ci ha detto che ci si dovrebbe giovare forse voleva dire addirittura beare - del fatto che si può fare tirocinio in uno studio di un certo livello, per cui basta poi far sapere che si è fatto pratica in quel tipo di studio che le porte si aprono. andando a vedere anche altri articoli della proposta di riforma, le porte non si apriranno perché ne sono state create di seconde, terze, quarte quinte, realizzando una vera e propria corsa ad ostacoli. questo ordine del giorno chiedono al Governo di assumere l'impegno: ad intervenire in merito alla regolamentazione del tirocinio, escludendo la previsione di oneri ingiustificati a carico del praticante; a prevedere lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario, introducendo a tal fine lauree abilitanti; ridurre la durata del tirocinio; a introdurre misure che riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo; a prevedere forme di sussidio (premi o borse di studio) al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale; prevedere e a valorizzare il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a quello effettuato presso gli studi legali privati ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, tenendo in considerazione anche, ad esempio, l'attività svolta presso gli uffici legali d'imprese, ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche e altre istituzioni in cui viene svolta attività legale. Paradossalmente, chi lavora per un Tribunale penale internazionale, per la Corte penale internazionale o per le Nazioni Unite deve ricominciare tutto daccapo. Infine, si impegna il Governo a rinnovare il meccansimo dei corsi di indirizzo professionale previsti obbligatoriamente ai sensi del presente disegno di legge, in maniera tale che la frequenza a tali corsi possa sostituire validamente il tirocinio diventandone parte integrante. Per questi motivi, chiediamo la votazione nominale con

ci occupammo dell'ordinamento giudiziario. Purtroppo, ciò che nuoce in questo momento ai fini della preparazione dei giovani sono le nostre università,

tutte le ragioni esposte in questi ordini del giorno sono più che fondate, relativamente alla circostanza che in questo modo non si favoriscono i giovani e che si creerà una sorta di casta chiusa, perché alla professione forense potranno accedere

corso di formazione per le professioni forensi che parificava la pratica fatta presso gli studi legali a quella svolta presso i magistrati. Forse la conflittualità che si è venuta a creare e che si sta creando tra magistratura e avvocatura dipende anche da questa pessima conoscenza. che uno dei nostri Padri costituenti disse a tale proposito che sarebbe stato opportuno che gli avvocati e i magistrati si scambiassero addirittura le loro funzioni. Invece, in questo ordinamento giudiziario vediamo che tutto ciò viene eliminato e che si chiude e si polarizza sempre la formazione esclusivamente sugli studi legali, fatto

Signora Presidente, l'emendamento 1.200 sarà da me ritirato: so che la senatrice Alberti Casellati ed il relatore sono dell'opinione di seguire un altro tracciato rispetto a quello che l'emendamento propone. Tengo a solo a dire due parole sulla via che era qui prefigurata: da una parte riconsegnare in tutto e per tutto al Ministro della giustizia, che ne ha la vigilanza, il compito, attraverso i regolamenti e la normazione secondaria, di dare attuazione alla legge;

a monte, attraverso la consultazione con il Consiglio nazionale forense e le più rappresentative associazioni di avvocati; a valle, attraverso un doppio controllo parlamentare da parte delle Commissioni permanenti. Tuttavia, come le ho anticipato,

se il relatore e il Governo riterranno che potranno essere utili e funzionali al risultato finale saranno accolti, altrimenti saranno destinati all'accantonamento definitivo. l'emendamento 1.201, abuso in questo momento della pazienza dei colleghi per fare una considerazione che non ripeterò poi più avanti in relazione ad altri emendamenti di uguale tipo. Sono forse delle puntigliosità, e me ne scuso, tuttavia ho ritenuto opportuno che un lavoro operoso, laborioso e attento su questo testo per farlo risultare il migliore possibile dovesse portare anche a questo tipo di emendamenti. Sono persuaso, signora Presidente, che i principi della Costituzione si rispettano senza bisogno di scriverli in una legge; credo invece che in una legge si possa oggettivamente scrivere che la stessa è in attuazione

mirano a rimuovere il vocabolo "imponendo" sostituendolo con il vocabolo "prescrivendo". Anche in questo caso, signora Presidente, converrà con me sul fatto che si tratta di una questione di modesto livello. Credo tuttavia che la legge non debba e non possa imporre mai alcunché: la legge prescrive. Si tratta di una di quelle ipertrofie retoriche, che forse sono state da sempre una caratteristica dell'eloquio dell'avvocato e che, secondo me, non hanno più necessità di essere. Vorrei che questo tipo di retorica fosse consegnata allo stereotipo dell'avvocatura e non entrasse nella nuova legge che la regolamenta.

accanto al rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, anche la dizione «e dei trattati internazionaliۛ».

procedure di infrazione alle norme europee e avanti alla Corte di giustizia europea siamo chiamati come Paese a rispondere di questi argomenti ormai da molti e molti anni. Ciò detto, visto che affrontiamo questo disegno di legge e in Assemblea possiamo fare tutte

Ricordo che l'Accordo GATS, sottoscritto nel 1986 da ben 117 Paesi a conclusione dell'Uruguay *Round* ed entrato in vigore in Italia nel 1995, prevede al primo articolo che lo che lo «scopo del Trattato è l'erogazione dei servizi in qualsiasi settore di attività, con la sola eccezione dei servizi necessari per l'esercizio dell'attività di Governo». La Commissione redattrice, che fu interpellata dalla Commissione consultiva degli ordini forensi europei, ribadì che «la professione legale è totalmente assimilata all'attività d'impresa, inclusa tra i servizi e soggetta, quindi, allo stesso processo di liberalizzazione» liberalizzazione» (questa parola magica che poi nella realtà e nel testo viene smentita dove è possibile). Veniva poi lasciata alla decisione delle singole autorità nazionali la possibilità di includere tra i servizi anche la difesa dei dei cittadini davanti alle Corti, mentre erano compresi gli altri aspetti della professione, in particolare la consulenza. Averla inclusa tra i servizi professionali nel quadro del commercio internazionale non rappresenta una *deminutio*, bensì il riconoscimento dell'importanza economica di questo settore e della sua dimensione internazionale. Tutti i servizi, al pari delle attività commerciali, sono inquadrati nel GATS, oggi WTO, nelle sessioni del quale cercano un coordinamento i problemi del commercio mondiale. La Corte di giustizia europea ha da tempo fissato il principio secondo cui «un'organizzazione professionale si comporta come un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Trattato - quando i membri del Consiglio sono esclusivamente rappresentanti dei professionisti e nessun organismo esterno può intervenire nella designazione dei membri, i quali non possono essere qualificati come esperti indipendenti e non sono obbligati da alcuna legge a prendere in considerazione (...) l'interesse generale». Peraltro, lo stesso articolo 85 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza. Le stesse decisioni della Corte di giustizia (casi Arduino e Cipolla) che hanno dichiarato l'ammissibilità delle tariffe, hanno motivato la decisione affermando che «le tariffe sono emanate dallo Stato che non può delegare ad operatori privati,

Secondo la Corte, inoltre, «gli ordini non hanno un ruolo pubblico e non tutelano interessi pubblici generali, ma sono associazioni di imprese che agiscono essenzialmente a fini privati e tutelano

chi visita i siti radicali, *Facebook* e quant'altro, ha fatto sì che o i collaboratori o gli stessi senatori in persona, tra cui

da quanto nella precedente legislatura fu concordato da parte di tutti gli ordini professionali con il Governo dell'epoca: dette vita al disegno di legge n. 2160 che riguardava le professioni intellettuali. Da quel disegno di legge noi abbiamo oggi scorporato la materia dell'avvocatura; ciò non toglie che alcuni principi generali siano perfettamente applicabili. Mi riferisco in particolare a quelle scelte innovative che vogliono evitare, nell'economia della conoscenza e dello sviluppo, una dipendenza degli avvocati da professionalità straniere (noi abbiamo infatti liberi professionisti particolarmente qualificati), impedendo di misurarsi nei mercati internazionali e, soprattutto, di sviluppare il merito dei giovani.

piuttosto un'identità proiettata nell'interesse dell'utenza, del libero mercato e, soprattutto, del futuro dei giovani. Infatti, soltanto una nuova e moderna ragion d'essere può giustificare il mantenimento del sistema ordinistico con il collaterale riconoscimento di associazioni professionali, sempre che rispondano agli interessi generali della prospettiva dell'utenza e della necessità di riconoscere un libero accesso ai giovani, sia pure con le dovute cautele per assicurare che il merito venga riconosciuto e che questo determini una selezione che successivamente il mercato produrrà nell'ambito dell'esercizio della professione. L'idea è quindi quella di dettare una disciplina di base a carattere generale, che in passato veniva lasciata ai decreti legislativi da approvare, e che oggi noi riteniamo debba invece essere approvata con regolamento del Ministro della giustizia (visto che è stata diversamente configurata la proposta di legge), purché vengano sentiti una serie di organismi e istituzioni che possano garantire al Ministro una consulenza sui temi di interesse. Mi riferisco, in particolare, alla necessità di sentire il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell'Ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative

come l'organo che avrebbe dovuto individuare le associazioni maggiormente rappresentative) e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di competenza. Inoltre, il Ministro può acquisire il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della giustizia. Comunque, non potendosi

le professionalità e l'associazionismo di vario genere e può interpellare anche tale Autorità per i profili di carattere economico e sociale e per le conseguenti ricadute. Tutto questo deve servire a garantire, attraverso il sistema ordinistico, la libertà di concorrenza dei professionisti, nonché il libero ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. prevede, come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio

ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni, il che è in linea anche con il parere della 5a Commissione. Tutto questo troverà sviluppo successivo nelle norme a favore dei giovani meritevoli e per la selezione del mercato anche attraverso la possibilità di prevedere una delega al Governo per l'istituzione di lauree abilitanti direttamente all'esercizio della professione.

colleghi, uno dei problemi più delicati nella regolamentazione delle libere professioni, direi forse il problema cruciale, è costituito da una gravissima asimmetria informativa tra il libero professionista e il cliente (o paziente, quando si tratta di un medico) non soltanto circa la qualità della prestazione che viene svolta ma talvolta addirittura circa l'oggetto della prestazione che deve essere svolta. Il professionista per definizione è quello che se ne intende, che sa; il cliente, invece, non sa. Questa situazione determina in numerose in numerose situazioni un conflitto d'interessi grave tra professionista e cliente. Il professionista si trova a poter scegliere tra diverse strade; diverse strade; e può accadere che quella più vantaggiosa per il cliente non sia quella più vantaggiosa per il professionista, nel nostro caso per l'avvocato.

il proprio patrono. Noi dobbiamo risolvere questo problema. L'Ordine degli avvocati deve fornire, nelle forme adeguate, questo servizio, che è la funzione principale che deve essere svolta dall'Ordine: non contro gli avvocati, ma nell'interesse del loro prestigio e della loro affidabilità.

in funzione di un controllo altrimenti impossibile. Nel panorama internazionale esistono diverse esperienze di questo genere. In funzione delle considerazioni svolte, abbiamo presentato l'emendamento 1.204

cioè di promuovere «in ogni forma possibile, il superamento dell'asimmetria informativa tra avvocato e cliente attuale e potenziale circa la qualità, i contenuti specifici e i possibili esiti della prestazione professionale».

Se non vogliamo farlo in questa maniera, facciamolo in un'altra: proponeteci qualcosa di diverso. Ma, badate bene, se questa legge non affronta e risolve questo problema,

Se poi decidiamo di non considerare la professione forense come assimilata ad un'attività d'impresa che sottosta al processo di liberalizzazione e decidiamo altresì che una libera professione in realtà

non possiamo alzare dei muri, tant'è che noi, nonostante l'elevato numero di avvocati presenti in Italia - elevatissimo come voi stessi ci dite - in realtà poi importiamo la consulenza legale. Noi impediamo la pubblicità agli studi

consultare gli Uffici. Per cortesia!

finestra"). Onorevoli senatori, vi è stata una situazione un po' complicata.

a tutela degli interessi della collettività, che devono essere - certo - contemperati con gli interessi economici e professionali degli avvocati. Su questo punto dobbiamo compiere una scelta che ci accompagnerà

della difesa e della tutela dei diritti; *d)* tutela l'affidamento della collettività e della clientela, imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale.

(...), promuovendo l'interesse del cliente in tutti i casi in cui si determinino conflitti di interesse tra lo stesso e l'avvocato». Non capisco questo emendamento: che significa «promuovere l'interesse del cliente nel conflitto tra

è contrario perché la Costituzione viene attuata. Quindi, è possibile usare l'espressione «nel rispetto di una Costituzione attuata»: questa affermazione mi lascia sperare per quello che sto per dire. Questa è una riforma necessaria e urgente, perché da 75 anni il Paese l'attende. In questi giorni, e mai come in questi giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche suoi validi rappresentanti e collaboratori, ci ricordano che la maggioranza è disposta ad attuare le riforme d'accordo con l'opposizione. Bene, io ribadisco che questa riforma, che arriva con 75 anni di ritardo, è una riforma necessaria, indispensabile e che mai come questa volta l'opposizione è disponibile disponibile e pronta a collaborare. E lo fa attraverso emendamenti. Questo è un emendamento, signora Sottosegretario, che dovrebbe essere attuato perché, come lei dice, è pura Costituzione. Noi modifichiamo l'ordinamento forense perché l'Italia ha una pletora di avvocati, un numero rilevante ed esorbitante di avvocati, spesso non all'altezza e con difficoltà enormi sul piano funzionale della giustizia. Dobbiamo dare al Paese un nuovo tipo di avvocato: un avvocato che sia in grado di attuare la Costituzione. Che facciamo, colleghi della maggioranza? Vogliamo forse chiedere ai 300.000 avvocati in carica di modificare di modificare la loro cultura, di adattarsi alle nuove esigenze di tipo internazionale, in quanto parliamo di diritto, ma anche di tipo concettuale e operativo nell'ambito del processo? Oppure, con la riforma noi puntiamo al futuro,

perché? Perché, signor relatore, probabilmente lei ha pensato che avrebbe comportato un onere. Ebbene, il puntuale richiamo della 5a Commissione ha trovato una puntuale risposta da parte nostra. Penso che molti di voi - scusate, non vorrei offendervi - non sappiano cosa stanno bocciando. È qualcosa di buon senso, qualcosa di corretto, qualcosa che punta a dare al Paese nuovi avvocati, rispettando, signora Sottosegretario, la Costituzione, nella parte in cui dice che tutti sono uguali e che tutti devono avere pari opportunità nel lavoro. Ma allora, che facciamo, una selezione per censo, censo, una selezione per potenza nell'ambito del sistema sociale? Oggi, per accedere ad uno studio professionale degno di questo nome e che dia garanzie per il futuro non bisogna essere un *quisque de* *populo*: bisogna avere delle garanzie sociali ed economiche. Per essere migliori di quello che oggi offre il Paese c'è bisogno di una preparazione culturale e professionale: e chi la può garantire a questa fascia di popolo, che sempre più

- e non ho sentito nessuno di voi che si sia alzato per dire che questo emendamento è fallace e che non è degno di essere applicato - voi non sapete che state bocciando la Costituzione. Noi chiediamo il rispetto per i giovani, le nuove generazioni, il futuro del Paese! Non c'è demagogia, non c'è posizione di sinistra o di destra: c'è semplicemente la volontà di dare all'avvocatura una dimensione nuova, nel rispetto dei principi costituzionali. Vi chiediamo pertanto di ragionare e di votare sì a questo emendamento.

e produce una situazione di totale caos, che poi è quella che già stiamo vivendo. Collega Maritati, se lei va sul sito Internet del CEPU troverà che oggi basta andare in Spagna a sostenere un esamino di omologazione della laurea italiana,

del PD in quella sede. Oggi mi accorgo che, invece, il Partito Democratico promuove una professione che è ormai equiparata ad un'attività di impresa e che quindi, come tale, deve essere garantita a tutti, senza nessuna forma di restrizione volta a preservare la qualità e la serietà professionale. Ecco i motivi per i quali non possiamo accettare un'impostazione di questo genere. Il diritto comunitario, se è diritto comunitario, rispettato da tutti i Paesi, può andar bene, ma non può accadere che la Spagna abbia una situazione tale per cui è sufficiente andare là, fare la *prueba* e si diventa *abogado* se il giorno dopo si viene in Italia ad esercitare la libera professione.

non ho capito se stiamo parlando dell'emendamento 1.208 o di un'altra cosa, perché l'intervento del collega Mazzatorta mi pare fosse eccentrico.

per modulare e creare delle griglie nell'accesso alla professione, considerato quello che sta avvenendo nel nostro Paese. Siamo secondi solo alla Grecia per numero di avvocati per abitante quindi, indubbiamente, si irrigidisce il sistema dell'accesso. Tuttavia, prevedere che questa rigidità nell'accesso non debba sacrificare quei giovani che hanno le qualità ma non le condizioni economiche per poter sviluppare la loro pratica, il loro tirocinio, la loro formazione

borse di studio o apposite fondazioni, utilizzando i fondi a disposizione o del Consiglio nazionale forense o dei singoli ordini territoriali, non mi sembra che rappresenti qualcosa di scandaloso. Si tratta di un'attenzione verso le nuove generazioni in una legge di impostazione generale. Penso

siccome la conosciamo e l'abbiamo apprezzata tante volte in quest'Aula, le vorrei chiedere di non comportarsi come se stessimo sventolando una muleta rossa.

compone il quadro di un modo assai moderno di intendere la professione forense. Qual è l'accezione classica e conservatrice della professione forense? È quella che prevede - come altre professioni liberali, naturalmente - una configurazione di tipo castale o corporativo, se volete, nella quale la stessa professione viene esercitata in un tramandarsi per generazioni, ostacolando l'ingresso dei nuovi talenti e dei nuovi meriti, in un Paese nel quale, peraltro, come lei sa molto meglio di me, l'indice della mobilità sociale è fermo. In questo contesto noi prevediamo, con questo emendamento, una serie di misure che agevolino l'ingresso e l'esercizio della professione a giovani dotati di talento e che non hanno alle spalle né lo studio di avvocato del padre o del nonno, né mezzi economici. Credo, quindi, che molto seria, peraltro fondata sul merito e sulla competenza (nella parte in cui si prevedono, per esempio, le borse di studio) e non fondata invece sulle sostanze economiche o sull'appartenenza familiare. Il fatto che, su suggerimento del senatore Lusi, sia stata eliminata la parola «libero» toglie ogni e qualunque equivoco in ordine al fatto che si voglia prevedere in Italia un ingresso e un esercizio della professione forense fuori da una valutazione del merito. Al contrario: i nostri emendamenti vanno tutti nella direzione di sottolineare la necessità che anche il filtro degli esami per l'ammissione alla professione sia tale

sia il riferimento al diritto comunitario ad intralciare una lettura chiara della norma, le dico due cose: innanzitutto, dovrete abituarvi al fatto che il diritto comunitario cominci a regolare ambiti sempre più vasti dell'agire della nostra società e del nostro sistema, siamo anche disponibili ad eliminare la parte che recita «garantisce l'ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario», proprio per evitare qualunque equivoco. Ci stiamo spendendo in questo modo perché riteniamo questo punto particolarmente qualificante e perché, qualora l'emendamento 1.208 non passasse, voteremo contro l'articolo 1

Voglio dire al relatore e al Presidente della Commissione giustizia che intendiamo affrontare questo tema

oltre ogni ragionevole e sensata esigenza di qualificazione della professione forense. Un conto è infatti che l'avvocato, che esercita una funzione costituzionale, cioè la tutela del diritto alla difesa,

e l'avvocatura presidino questo tipo di interesse; un altro conto è che, sotto la scusa della tutela di questo fondamentale diritto costituzionale, si chiuda l'accesso alla professione, lasciandolo solo a pochi privilegiati o a chi ha condizioni economiche tali da poter reggere un tirocinio che diventa anch'esso

un po' forsennati - lo hanno elaborato, nascondendo, dietro la tutela di un fondamentale diritto costituzionale, l'esigenza di evitare che nel settore dell'avvocatura ci sia concorrenza. allora che, se vogliamo ridare equilibrio intanto dal punto di vista dei principi che regolano questa materia, l'idea di attribuire all'Ordine anche il compito di favorire la qualità nelle giovani generazioni che vogliono accostarsi ad un'avvocatura nuova, moderna e più qualificata sia una questione di buonsenso che dovrebbe trovare tutti d'accordo, anziché chiusi nella difesa corporativa

con misure come la limitazione del riconoscimento dei titoli: dovremmo farlo invece attraverso un'iniziativa del Governo in sede comunitaria perché, sotto il profilo della tutela delle professioni, si faccia qualcosa in più.

obiettivamente ridicola e - lo dico con rispetto per i colleghi della Lega - anche in qualche modo in controtendenza rispetto alle pratiche federaliste di queste settimane e di questi giorni. Allora, per evitare che diventi motivo

Presidente, c'è un'ipotesi di riformulazione che, alla luce degli argomenti introdotti, mi pare possa essere presa in considerazione. Se la collega Della Monica ritiene di poter accedere alla nostra proposta, riformulerei l'articolo in questa maniera: «prevedere come compiti degli organi nazionali e territoriali anche l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare...»,

l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11».

Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori. Mi spiego in maniera molto sintetica. Questa materia - lo dico al relatore, al rappresentante del Governo e ai colleghi dell'opposizione - è straordinariamente tecnica e ovviamente affidata alla sensibilità particolare degli operatori della materia giuridica e giudiziaria: agli avvocati che sono presenti in quest'Aula e ai magistrati. La mia considerazione, da legislatore ordinario, è che l'andamento di questa normazione non stia portando da nessuna parte. Mi spiego: se l'articolo 1, che definisce i principi di questa legge, non trova una definizione - i colleghi del Partito Democratico hanno proposto nei fatti una formulazione alternativa indiretta

la minoranza a valutare se una legge che non riesce neppure a trovare l'intesa sul primo articolo non meriti un ulteriore approfondimento. Voglio dire, Presidente, che noi possiamo un esame di dettaglio di centinaia di emendamenti, destinati a recepire un aspetto anziché un altro ma, se volete la mia previsione, all'atto di fare una dichiarazione di voto sull'articolo 1, questa legge non andrà da nessuna parte, perché si sta procedendo in maniera disomogenea. Mi permetto di osservare che lo stesso emendamento che ha illustrato prima il collega Maritati contiene aspetti di dettaglio talmente penetranti sulla destinazione delle risorse degli ordini professionali, oltre che sulle modalità di apertura e chiusura della professione che ho la sensazione che si stia preparando un pasticcio.

la mia sensazione non è lontana da quella appena espressa dal senatore Rutelli. Premetto

di scelte particolari, attuative di queste finalità. Di talché si potrebbe anche ritenere che facilitare l'accesso alla professione forense da parte dei giovani aspiranti professionisti si realizzi meglio con alcuni strumenti,

Presidente, non mi pare che stiamo facendo male. Stiamo facendo bene e stiamo trattando l'articolo 1 che è l'articolo essenziale, fondamentale: è quello che detta i principi. Voglio rammentare che sui principi, sugli aspetti fondamentali dell'esigenza di innovare eravamo tutti d'accordo, salvo poi introdurre una serie di modifiche che incidono in maniera marginale, ma che certamente non ledono il principio ispiratore dell'articolo 1. In considerazione di ciò ritengo quindi che sussistono tutte le condizioni per andare avanti. Se per avventura un emendamento dovesse essere meritevole di un'attenzione particolare, così come è accaduto, il dibattito in Aula consentirà una valutazione la più opportuna possibile. di versare in una condizione un po' imbarazzante. Ho condiviso il lavoro fatto dal relatore, senatore Valentino, nel Comitato ristretto; ho condiviso il suo sforzo per arrivare ad un testo su una materia estremamente delicata,

ma noi sappiamo benissimo, per l'esperienza maturata in questi anni, che è cosa diversa affrontare alcuni temi nel dibattito nella sede propria, nella Commissione di competenza. Forse è opportuno, onorevole collega relatore, onorevole Presidente della Commissione,

non avventurarci in un dibattito in Aula, purtroppo, inevitabilmente condizionato dalle presenze in Aula, presenze in Aula, così facendo prevalere valutazioni politiche rispetto ai contenuti tecnici di un provvedimento: qualora infatti si colga la possibilità di una momentanea assenza della maggioranza si potrebbero votare cose di cui tecnicamente non si è convinti. Allora, considerata la delicatezza della materia

senatore D'Alia.

un po' fuori di logica la circostanza che non si accetti si accetti che un principio introdotto, quello della libertà di concorrenza dei professionisti, debba essere tutelato dall'Ordine. Ma se l'Ordine non deve garantire che non vi sia una concorrenza sleale tra avvocati, di che cosa si deve occupare? Ed è ancor più grave negare l'affermazione esplicita di questo principio, chiedendone la eliminazione dal testo dell'emendamento. Se dobbiamo discutere di tali questioni,

Signora Presidente, con lo stesso rispetto e atteggiamento costruttivo che mi pare stia emergendo da più parti nell'Assemblea,

il gratuito patrocinio, cioè l'esercizio effettivo del diritto di difesa d'ufficio, l'accesso dall'università alla professione, che poi è il vero problema che conoscono le migliaia di giovani avvocati italiani, cioè quante persone, in relazione alla riforma dell'università, effettivamente possano accedere alla professione ed alle diverse articolazioni nel campo giuridico

sull'articolo 1, cioè sui suoi principi, non ci si possa addentrare in una attività emendativa di dettaglio. Come minimo, la maggioranza, e auspicabilmente le opposizioni, dovrebbero convenire sui principi di questa normativa, dopodiché si potrà entrare nella discussione che riguarda

sollevai la questione di un provvedimento di questo genere (peraltro - riflettete colleghi! - anche capofila, sotto il profilo dei principi che verranno con esso disegnati, della riforma delle professioni che il Governo pare intenzionato ad affrontare di seguito). Un provvedimento così, gravato di La ragionevolezza La ragionevolezza non è stata premiata ieri mattina. Mi pare che la discussione di oggi testimoni della necessità di tornare in Commissione. Senza però che ci nascondiamo dietro ad un dito, Presidente: qui quello su cui ci si scontra non è soltanto la normativa di dettaglio, non sono i 730 emendamenti, tutti corrosivi di

quale sia l'ordinamento forense utile all'Italia oggi; si scontrano due diverse concezioni, molto chiaramente, già sull'articolo 1 da questo primo emendamento presentato.

anche della concorrenza, nelle mani del Consiglio nazionale forense, cioè del sistema: chiamiamolo casta o corporazione, solo per intenderci, fuori da ogni volontà

anche sotto questo profilo, al nostro Paese di competere. È fin troppo chiaro. Questo ovviamente matura un giudizio politico sulla maggioranza e sull'operazione di conservazione - altro che modernizzazione! - che sta facendo in uno dei settori più importanti della vita del Paese. C'è quindi un'opposizione - e sono felice che si parli la stessa lingua tra forze di opposizione che pure hanno storia e cultura politica assai diverse - che vuole consegnare all'Italia un sistema professionale (oggi con gli avvocati, domani con i commercialisti o con i farmacisti o con i notai) che sia assolutamente non solo aderente a quello che avviene nel panorama europeo, ma anche tale da smontare il potere della successione ereditaria e delle corporazioni. Sono da consegnare nelle mani delle giovani generazioni nuovi strumenti ed opportunità per la loro crescita e per la crescita del Paese. Il punto è questo. È un punto di principio. È un punto politico. Ed è, purtroppo, il punto politico sul quale io credo saremo chiamati anche a tornare in Commissione, altrimenti quello che potrà scaturire da un testo gravato da 730 emendamenti, con votazioni che, come abbiamo visto poc'anzi, possono essere anche del tutto casuali, sarà probabilmente un obbrobrio nel quale nessuno di noi vorrà riconoscersi.

Naturalmente i meccanismi emendativi cercheranno di renderla ancor più aderente alle esigenze della società e dell'avvocatura. È per questo che siamo qui a discuterne. Onorevoli colleghi, se ogni volta il numero degli emendamenti dovesse impressionare l'Aula e imporre

l'avvocatura italiana reclama e sulla quale tutta era d'accordo.

si scontra con la storia in Commissione di questo provvedimento. Voglio ricordare che il Comitato ristretto aveva lavorato per mesi trovando un'ampia condivisione su certe scelte, ma poi ci si trovò in Commissione di fronte al fatto che lo stesso rappresentante dell'opposizione aveva firmato degli emendamenti contrari alla sua stessa decisione resa in sede di Comitato ristretto. Poi, non comprendo perché, quando si afferma che l'Assemblea è libera e che i senatori devono decidere secondo coscienza,

si prevede che «la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta

perché mirano a deparlamentarizzare ulteriormente il processo di legislazione. Su questo non sono personalmente d'accordo. Per quanto riguarda l'emendamento

l'opportunità di non privare il Governo, attraverso la soppressione del comma 6, della possibilità di introdurre norme integrative e correttive In sintesi, con tutto il rispetto ed il riguardo possibili e - come si usa dire - in maniera sommessa, suggerisco al relatore e al rappresentante del Governo di modificare il proprio parere con riferimento all'emendamento 1.230,

questo emendamento serve a ristabilire un punto di equilibrio, un punto di equilibrio, nel senso che il Parlamento, il Governo ed in particolar modo il Ministro della giustizia, che ha il compito di vigilare e discutere con gli ordini professionali ed il mondo delle professioni, non può e non deve scrivere le proprie norme sotto dettatura di nessuno. Questo vale per il Consiglio superiore della magistratura e per l'Associazione nazionale magistrati ma, per chi sostiene il principio della parità e della pari dignità tra difesa e accusa, vale anche per gli organi rappresentativi dell'avvocatura; altrimenti c'è qualcosa che non funziona. Pertanto, se così è, tutti i regolamenti di attuazione della normativa sulla professione forense non possono essere preventivamente scritti sotto dettatura del Consiglio nazionale forense. del Consiglio nazionale forense. Quest'ultimo, insieme agli Ordini professionali e al sistema rappresentativo dell'avvocatura, deve contribuire, ma non può essere il soggetto che si sostituisce al Parlamento e al Ministro nella stesura e nella disciplina di questi aspetti. aspetti. Altrimenti, cari colleghi della maggioranza, se si fa passare questo principio nella legge sulla professione forense, a maggior ragione lo stesso principio lo dovrete invocare con riferimento al ruolo della magistratura nel rapporto con le attività che svolge e con l'attività normativa del Parlamento e del Governo.

si riteneva di non dover aumentare il numero di anni entro i quali passare ad una serie di ulteriori regolamenti. Il giudizio favorevole su questo emendamento è rafforzato anche dalla risposta che ha dato ad un certo punto il relatore, dicendo che questo provedimento impone, impone, impone... In effetti, esso impone tante cose; però, bisogna vedere chi è che detta queste imposizioni. Egli ha anche detto che l'avvocatura italiana reclama questo tipo di riforma. Mi è stata poco fa girata per *e-mail* - la leggo - la dichiarazione dell'avvocato Renato Borzone, vicepresidente dell'Unione camere penali italiane, che si riferisce in particolare ai 180 (più 180, a questo punto) emendamenti che la delegazione radicale avrebbe presentato di riforma della controriforma,

«In questi ultimi giorni le iniziative della giunta per tenere in piedi la battaglia per la dignità e la qualità dell'avvocatura hanno raggiunto un impegno parossistico. Più di così non si poteva fare, e non lo si dice per difendere se stessi. Tutto il resto, quel che succederà da domani appartiene forse - abbiamo cercato di evitare che sia così - all'area dell'incontrollabile ed a quella - speriamo non insufficiente - del razionalmente possibile. L'ultimo attentato - addirittura - che proviene dalla stessa maggioranza è la posizione della Commissione bilancio: un gioco delle tre carte di una politica inconsistente, senza valori e senza ideali. Credo si debba vendere cara la pelle e, se sarà necessario, far vedere di che pasta è fatta l'avvocatura penale a partire dal prossimo Consiglio dell'8 maggio. Certo, una grande, immensa amarezza è rappresentata tra l'altro dalla deriva radicale, movimento ormai consegnato alla logica della sopravvivenza spicciola, anche economica, e della demagogia da quattro soldi. Che tristezza e che dolore assistere a tutto questo. Ma non è detta l'ultima parola. La sola battaglia persa è quella che non si combatte». è quella che non possono combattere tutti coloro i quali non fanno parte dell'armata, dell'esercito dell'avvocatura italiana adesso. Si vuole, con questo disegno di legge, ancora una volta non soltanto alzare tutte le palizzate che sono state messe in evidenza nella discussione generale e nell'argomentazione a favore dei vari emendamenti che caratterizzano già quest'articolo 1, ma addirittura si vuole fare accompagnare qualsiasi tipo di ulteriore decisione dal parere del CNF. Ripeto che in questo disegno di legge

Ma non garantisce nessun tipo di libertà individuale. Quando questo avviene da parte dell'avvocatura italiana, credo che ci sia da preoccuparsi ben oltre il merito del disegno di legge in questione. Quindi, anch'io dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento

il senatore D'Alia legge il comma 3 dell'articolo 1 in maniera che non si può francamente accettare: lo dico col massimo rispetto. Dice il senatore D'Alia che il CNF non può dettare le proprie regole. Ma i Regolamenti vengono emanati dal Ministro della giustizia, previo parere,

si dovrà regolamentare. Non si preoccupi, senatore D'Alia: il CSM, com'è noto diffusamente, dà i pareri comunque, anche se non gli sono

emendamento può essere conseguente all'emendamento precedente con il quale si chiedeva che i regolamenti attuativi fossero emanati direttamente dal Ministero.

Senatrice Poretti, forse abbiamo testi diversi. Le posso far osservare che al comma 3 dell'articolo 1 è scritto che i pareri del CNF devono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta del pubblico ministero? Posso anche farle presente che l'emendamento 1.213, di cui stiamo trattando ed al quale preannuncio il voto contrario, diversamente da quanto lei dice, non prevede un termine? Quindi, vediamo di non fare demagogia su fatti che non sono nemmeno veri. C'è un termine di 90 giorni previsto al comma 3; non c'è un termine, in compenso, nell'emendamento che stiamo votando, ma c'è - ah sì, che gioia! - il parere del Consiglio superiore della magistratura. [LI

Si è molto disquisito sulle espressioni «previo parere» e «sentito». Ora, con questo emendamento, l'opinione del Consiglio nazionale forense diventa «sentita», però si eleva a parere quello del CSM. Mi sembra si sia data una graduazione a queste due espressioni, per cui il parere sarebbe più vincolante; e perché il Consiglio nazionale forense deve essere sentito e il CSM deve esprimere un parere? Tutte le perplessità che ho su questo tipo di strutturazione mi sembrano non condurre verso un voto favorevole, anche perché, lo ricordo, i regolamenti devono essere poi emanati dal Ministro della giustizia

**Il Senato non approva.**

Colleghi, per cortesia, ognuno voti per sé:

Chiediamo che vengano sostituite le parole «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le parole «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni». Conseguentemente, ci soffermiamo anche

di questo disegno di legge - di ridurre alcuni dei danni, che noi riteniamo essere gravi, che vengono imposti a chi da poco è presente sul mercato o a chi da poco si è costituito come associazione. Invitiamo, quindi, ad un voto favorevole

può sedersi o meno a dettare le regole. [LI

il secondo criterio perde la sua oggettività, perché introduce un momento valutativo e discrezionale

disomogeneo; ad un criterio oggettivo, che dovrebbe avere più forza, viene affiancato un criterio discrezionale che ha prevalenza sul criterio oggettivo e che, così

prevista che risulterebbe vincente sull'oggettività richiesta.

A questo punto mi fido sempre meno. Quali sono i problemi di *drafting* che vedremo dopo che abbiamo votato un testo? Visto che ne sono già stati accantonati due, accantoniamo anche questo emendamento! La fiducia è una cosa seria; avendo avuto a che fare con una fiducia mal riposta - pare di capire

e andiamo avanti a vedere stancamente tutti gli altri emendamenti: valutate voi! Io sono sempre contraria a sospendere le sedute, perché già il Senato lavora

Il problema che questi emendamenti affrontano è sostanzialmente quello del modo migliore con cui la legge, l'ordinamento e l'attività dell'Ordine forense possono garantire la qualità della prestazione dell'avvocato. Il primo comma del testo al nostro esame detta una norma che intenderebbe vietare l'esercizio dell'attività di assistenza legale a chi non la svolga in via abituale o prevalente.

di episodi, di casi anche particolarmente noti, di attività di difesa giudiziale svolta da soggetti

avvocati pensionati, che pur non svolgendo più la professione in via abituale hanno fatto eccezione in singole occasioni, oppure casi di docenti universitari. Perché vietare vietare che la professione possa essere utilmente svolta anche da chi non la svolge più in modo abituale? Per altro verso

Invito tutti i colleghi a considerare che il divieto di svolgere attività di consulenza stragiudiziale a chi non sia iscritto all'albo non ha alcuna giustificazione né sul piano tecnico, né sul piano professionale. È pacifico che è consentito anche a chi non è iscritto all'albo svolgere attività di legale d'impresa, per esempio, in forma di lavoro subordinato;

nel momento in cui va in pensione, continuare a svolgere quell'attività, mettere a frutto le sue competenze in forma di collaborazione autonoma continuativa? Mi spiegate per quale motivo ciò

di lavoro autonomo? Per quale motivo una società capogruppo non può mettere a disposizione delle società del gruppo la competenza in materia di diritto del lavoro, in materia di brevetti, in materia di diritto internazionale di un suo dirigente, o di un suo funzionario? funzionario? Su questa norma il testo che ci state proponendo si pone contro non soltanto l'orientamento dell'Unione europea e dell'*Antitrust*, ma anche di tutte, tutte, le associazioni imprenditoriali, le quali hanno preso una posizione molto netta contro questo divieto. L'unica spiegazione

Se qualcuno darà consulenza senza averne la competenza sarà l'informazione, la concorrenza a metterlo fuori mercato, in questo modo noi adottiamo un criterio di selezione che non corrisponde alla qualità e alla difesa dell'affidamento del cliente e della collettività.

perché noi, come successivamente chiarirà il senatore Galperti che interverrà su questo punto, riteniamo che possano essere iscritti all'albo non solo coloro che hanno superato l'esame di Stato, ma anche determinate categorie professionali che ne hanno i requisiti. Ricordo a tale riguardo, gli avvocati dello Stato, i professori universitari specializzati nelle materie giuridiche, i magistrati, che superano un esame ben diverso perché composto composto di tre prove scritte (un vero e proprio esame di Stato) per l'ingresso alla professione: esercitano l'attività e le funzioni, ma non hanno la competenza per iscriversi all'albo degli avvocati, quando loro stessi hanno formato la giurisprudenza a cui gli avvocati

Stiamo cercando di realizzare la riforma dell'accesso alla professione forense: se dobbiamo parlare dell'abolizione del titolo di studio di studio e della eliminazione dell'esame per l'accesso alla professione facciamolo, però diciamolo in maniera chiara. certo che il mio Gruppo non è favorevole ad una norma neocorporativa o fortemente corporativa;

e principale, altrimenti apriamo una serie di varchi che non controlliamo: non possiamo lasciare

Prego Visto però che non si degnano di intervenire in Aula, forse è il caso di dare una spiegazione del perché noi avevamo scritto quegli emendamenti e li abbiamo presentati, e anche i senatori Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva e Villari li hanno presentati: ringraziamo sempre che li abbiano, evidentemente almeno in una qualche fase della loro vita, condivisi e speriamo che poi vengano a sostenerli in Aula; altrimenti davvero fa

tutta la discussione e va a disciplinare la professione dell'avvocato. Su questo articolo abbiamo presentato diversi emendamenti,

nella direzione opposta. Quando al comma 3 dell'articolo 2 si stabilisce che «l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato»

tutto quel mondo che già fornisce un'assistenza stragiudiziale; mi riferisco ai sindacati, ai patronati, alle associazioni di consumatori e perfino ad

Dovrebbe certamente essere utile ripensare la figura dell'avvocato in chiave realmente libera ed autonoma, eliminando l'obbligo della abitualità dell'esercizio della professione. Si propone quindi anche di anticipare il momento in cui si può svolgere l'attività forense forense al momento del superamento dell'esame e non già all'iscrizione all'albo presso gli ordini. Crediamo debbano essere eliminate anche tutte le ipotesi di esclusiva che vorrebbero istituire

un parere o una consulenza. Per fortuna, come si è ripetuto, tutto ciò contrasta con gli obblighi internazionali e in qualche modo dovrà essere riformulato integralmente, se non qui, in sede di esame degli emendamenti, successivamente, quando verrà la direttiva comunitaria n. 22 del 2002 relativa al servizio universale obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione procedure extragiudiziali per l'esame delle controversie. Se la Se la risoluzione extragiudiziale è trasparente, semplice e poco costosa, la direttiva consente una risoluzione obbligatoria delle controversie. È chiaro che se ci si dovesse rivolgere ad un legale verrebbe meno la possibilità

ho deciso di lasciare il Gruppo del Partito Democratico e di iscrivermi al Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie. La mia decisione è stata condivisa e supportata all'unanimità dagli organi del Movimento dei Repubblicani Europei, che ho qui l'onore di rappresentare. La scelta del Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie non modifica la mia collocazione di schieramento, che è di ferma opposizione nei confronti di questo Governo, ma intende privilegiare - come è nella tradizione dei repubblicani - le questioni di contenuto e quindi valutare autonomamente nel merito e nei fatti concreti quale debba essere il giudizio sui provvedimenti che il Senato sarà chiamato a discutere. La decisione di lasciare il Gruppo del Partito Democratico viene da lontano. Nel corso di questi anni è apparso sempre più chiaro che il PD, che ha voluto escludere dall'atto fondativo la componente laica repubblicana, si è risolto nell'incontro di vertice tra un'area del mondo cattolico e la vecchia tradizione marxista. La tenaglia tra ex DS ed ex DL esclude proprio quelle culture e quella visione politica che si riassumono nella democrazia liberale e che sono alla base delle moderne società occidentali. In queste condizioni, dopo tante e sofferte battaglie, ho deciso di riprendere autonomamente la battaglia del Movimento dei Repubblicani Europei per continuare l'impegno per la democrazia e la difesa dei suoi valori fondanti che oggi sono in pericolo. C'è, però, anche un'altra ragione che mi spinge in questa direzione. Il sistema bipolare, divenuto bipartitico di fatto, così come costruito in Italia produce solo guasti endemici ed un'endemica inadeguatezza della politica nella sua esigenza di fondo che è quella di confrontarsi con i problemi del Paese. Sono in molti oggi, nell'uno e nell'altro schieramento, che ne vanno prendendo atto. Allora, è venuto il momento di superare questa visione miope e costrittiva della vita politica, di tornare a guardare e a collegarsi con le grandi famiglie della tradizione europea, di ridare identità e ruoli definiti ai partiti che cercano il consenso, si candidano a governare, forti di cultura e di tradizione democratica. In quest'ottica continuerà il mio impegno di parlamentare e di dirigente politico. Al Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie darò il mio personale contributo per costruire e rafforzare una delle grandi famiglie europee, nella quale da sempre mi riconosco: la famiglia della liberaldemocrazia. Il bipolarismo all'italiana ne ha mortificato la presenza, nel centrodestra come nel centrosinistra; superare lo schema bipolare significa anche creare le condizioni per il superamento di questo bipartitismo di fatto, perché la democrazia liberale possa tornare ad occupare il suo spazio, a vivere e ad esistere in autonomia, a lavorare per modernizzare il Paese. È l'obiettivo per cui lavorerò, assieme ai Repubblicani europei, in una presto ritrovata unità repubblicana.

si sono succedute varie ricostruzioni giornalistiche, alcune esatte e altre un po' faziose, rispetto ad avvenimenti e vicende che si sono verificati a Reggio Calabria in seguito all'arresto di un pericoloso latitante.

Diventa però difficile dare tutto questo spazio ad una cinquantina di familiari e parenti dell'arrestato e non dare lo spazio che meritano centinaia di persone che, appena venute a conoscenza dell'accaduto, si sono riversate davanti alla questura. Insomma, c'è una Calabria che non tace, che non sta in silenzio, che scende anche in piazza quando arriva il momento, ed è a quella Calabria che ci rivolgiamo con un ringraziamento. È una Calabria fatta di gente perbene, onesta, laboriosa,

di Milano, hanno dovuto travasare il contenuto di due ferrocisterne, contenenti ciascuna circa 40.000 chilogrammi di GPL che non sono risultati a norma. Il convoglio era in transito sullo stesso tragitto Trecate-Gricignano i convogli che hanno causato la strage di Viareggio. Meno male che i controlli messi in atto dall'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie hanno funzionato. Ma quando si capirà che bisogna far cessare sul nostro territorio il transito di queste cisterne *killer*? Lo sapete che il tratto Trecate-Gricignano attraversa ben 120 Comuni, tra cui Novara, Genova, La Spezia, le mitiche Cinque Terre, Massa, Roma, Latina? Sono tutti Comuni a rischio. Quello che è successo a Viareggio poteva succedere in ognuno di questi Comuni. Ma lo sapete che a dieci mesi dalla strage, con quattro inchieste avviate, ancora non si conoscono i nomi, non dico dei colpevoli, ma degli indagati? Vi rendete conto che un altro disastro è stato evitato solo grazie al sistema di controlli avviato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, questa Agenzia deve essere messa in grado di funzionare ed essere dotata di mezzi e di personale? Ragazzi, in questi 120 Comuni ci siamo tutti noi: abbiamo delle responsabilità verso i nostri territori. Ma cosa si deve fare per far cessare il transito di questi convogli? Che cosa dobbiamo fare? Altrimenti, altro che registro degli indagati! I colpevoli siamo noi! Ora basta!

L'Europa sta bruciando: la crisi greca, le responsabilità di questi "bankster", i banchieri di affari che condizionano le politiche, si comprano il silenzio dei Governi. Voglio ricordare che Goldman Sachs è alla sbarra davanti al Senato americano e che queste battaglie le porto avanti già da prima che mettessi piede in quest'Aula, combattendo queste banche di affari che speculano per avidità di guadagno, la collusione delle autorità monetarie e delle agenzie di *rating*. Andiamo a vedere chi c'è dietro Standard and Poor's,

c'è Citigroup. Chi c'è dietro Moody's? C'è J.P. Morgan. Quelli che hanno emesso questa montagna di derivati finanziari. Ho presentato Ho presentato tantissime interrogazioni parlamentari. Abbiamo approvato una mozione all'unanimità su una nuova Bretton Woods. È strano questo silenzio rispetto ad una questione che riguarda la vita dei popoli, la sovranità degli Stati. Il presidente Baldassarri della Commissione finanze sa che spesso denunciamo tali questioni. Signora Presidente, mi consenta di terminare l'intervento, perché non è possibile che ci siano questi banchieri che fanno quello che vogliono: il gioco sporco, ossia queste queste grandissime speculazioni. Oggi, un economista che si chiama Paul Krugman ha denunciato lo stesso conflitto d'interesse di queste grandi banche di affari e ha agenzie di *rating*, quelle che hanno elargito valutazioni di tripla A, il massimo possibile, ad *asset* di dubbio valore, per miliardi di dollari: quasi tutti questi giudizi si sono rivelati tossici. Non si tratta di un'esagerazione. Il *rating* del 93 per cento delle obbligazioni garantite da *subprime*

bisogna occuparsi di queste questioni, perché - lo ripeto - l'Europa brucia ed i banchieri si elargiscono prebende con *stock options*; l'Europa brucia e bruciano i posti di lavoro. E i Governi democratici, spesso condizionati da questi bankster - metà banchieri, metà *gangster* - con la prevalenza dei secondi che agiscono molto peggio di Al Capone,

Non è più possibile tollerare questo; questa speculazione si riverbera sulla povera gente, che poi paga il conto; i banchieri brindano a *champagne* con 5-6 milioni di euro - come Profumo - di *stock options*.

comportante spesa, ai sensi dei precedenti periodi, può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Sempre secondo la legge, in caso di violazione la RAI e gli stessi consulenti sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a 10 volte l'ammontare della somma illegittimamente